si apre un nuovo capitolo per i diritti dei figli naturali e si cominciano ad apportare alcune lievi ma significative modifiche al diritto di famiglia. Finalmente, l'esercizio della potestà genitoriale per i figli naturali spetterà ad entrambi i genitori anche dopo la separazione, ovvero con l'interruzione della loro convivenza, perché, se entrambi i genitori hanno riconosciuto il figlio, è giusto che entrambi se ne prendano cura ed esercitino la potestà. Inoltre, si specificano meglio le competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni.

Si tratta di un provvedimento all'apparenza semplice, ma dall'alta valenza politica, che segna un'importante pagina di storia parlamentare poiché, di fatto, serve a sanare un *vulnus* rispetto ad un'innaturale ed illogica dicotomia, eticamente inaccettabile, con riguardo alla disparità di trattamento dei figli legittimi rispetto a quelli naturali, contrastante con il comune sentire della nostra società che si evolve. Il sacrosanto principio della bigenitorialità, alla base della legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso, da cui anche questo provvedimento deriva, è inderogabile e non ammette distinzioni e discriminazioni di sorta: per questo si applicherà anche ai figli riconosciuti nati al di fuori del matrimonio. In oltre, con questo testo, si comincia finalmente ad eliminare l'ingiustificata duplicazione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, fondata unicamente sulla diversa qualificazione

Si tratta di un primo e importante passo in avanti verso il perfezionamento di un ordinamento che si incentri sempre di più sul cardine essenziale della tutela del minore, in cui l'interesse predominante sia sempre quello dei figli. Partiamo da un presupposto inderogabile che è quello per il quale, in caso di separazione dei genitori, il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con l'ascendente e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. È evidente che l'introduzione del principio di *favor* della condivisione dell'affidamento, anche in caso di separazione personale, rende anacronistica la disciplina recata dal secondo comma dell'articolo 317-*bis* ordine all'attribuzione della potestà sul figlio naturale riconosciuto in caso di non convivenza dei genitori che abbiano entrambi effettuato il riconoscimento. Tuttavia, pur essendo anacronistica, la norma non è stata modificata o abrogata dalla legge n. 54 del 2006. Ciò ha determinato, in tutti questi anni, uno stato di incertezza nella giurisprudenza che la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007, ha risolto considerando vigente l'articolo 317-*bis*. Di conseguenza, il tribunale dei minorenni è tuttora competente in materia di affidamento dei figli naturali, essendo, per l'appunto, l'articolo 317-*bis* tra quelli richiamati dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile che fissa la competenza del tribunale per i minorenni. Per i figli naturali quindi permane, da un lato, una normativa che non è ispirata al principio dell'affidamento condiviso e, dall'altro, un sistema barocco di competenze per il quale è il tribunale dei minorenni a decidere dell'affidamento, mentre il tribunale ordinario si pronuncia sulle questioni economiche relative al mantenimento dei figli stessi (articoli 248 e 261 del codice civile). Il testo che ci accingiamo a discutere e a votare oggi è l'unificazione di due disegni di legge che si proponevano di risolvere le incongruenze relative alla disciplina giuridica della condizione dei figli naturali.

concernente le decisioni del giudice e le relative modalità in materia di esercizio della potestà dei genitori, che trova ancora applicazione relativamente ai figli naturali. L'articolo 3 novella l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ridefinendo la competenza del tribunale dei minori in sede civile. Con questo testo dunque, lo ribadisco, si comincia ad eliminare finalmente l'ingiustificata duplicazione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, fondata unicamente sulla diversa qualificazione di uno dei soggetti coinvolti quale figlio nato all'interno o al di fuori del matrimonio. Non solo: come relatore propongo un emendamento con cui si pone rimedio ad un vuoto normativo, modificando l'articolo 276 del codice civile sulla legittimazione passiva. Oggi, infatti, in caso di morte del genitore vengono considerati legittimati passivi i suoi eredi, ma quando vengono meno anche gli eredi diventa impossibile individuare altri legittimati passivi all'azione di riconoscimento del genitore. Con questo emendamento, invece, il figlio, in mancanza del presunto padre o della presunta madre, dovrà proporre l'azione in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

*relatrice*. Ricordando nuovamente all'Assemblea che questo disegno di legge porta la firma del presidente del Berselli e di tutti i Capigruppo della Commissione giustizia e che in tale sede è stato approvato all'unanimità, auspico che lo stesso possa avvenire in Aula quest'oggi, alla luce dell'importanza della materia trattata e del fatto che il provvedimento rappresenta un primo passo importante che apre la strada ad ogni possibile ulteriore provvedimento verso quella che io chiamo, in maniera poco formale, la legge Filomena Marturano. finestra"). Comunico che è stata presentata la questione sospensiva

nel sistema giuridico delle relazioni familiari e dei diritti dei minori le cose devono restare come sono o c'è bisogno di una riforma? Non è una domanda retorica. C'è assolutamente e urgente bisogno di una riforma. Nel nostro Paese abbiamo avuto alcuni momenti alti, nei quali le diverse tradizioni politiche e culturali hanno operato una sintesi feconda, cogliendo la domanda di giustizia e di maggiori diritti delle cittadine e dei cittadini. Pensiamo alla fase costituente e alla grande riforma del diritto di famiglia del '75. Oggi, i cambiamenti nella società e nella famiglia chiedono di rispondere alla domanda di giustizia con lungimiranza, senso di responsabilità e coraggio nella sfida della sintesi. Noi siamo pronti per una vera riforma. Una grande riforma che metta al centro la persona umana, a partire dal bambino e le sue relazioni. Basta con la frammentazione delle competenze tra giudici diversi; basta con l'assenza delle garanzie del giusto processo nei procedimenti minorili e di famiglia; basta con le diseguaglianze dei diritti, riconosciuti o meno, in situazioni sostanzialmente identiche; basta con le diseguaglianze tra bambini a seconda se i genitori decidano di sposarsi o meno. I figli naturali, per la legge, non hanno nonni o altri parenti. Basta con la diversità dei riti processuali e delle connesse garanzie; basta con giudici lontani e non prossimi ai cittadini. In questo ambito, cosa deve fare una riforma per essere chiamata tale? Intanto deve essere una riforma organica e di sistema. La persona e le sue relazioni devono essere poste al centro della riunificazione delle competenze e della riorganizzazione del sistema processuale e sostanziale. Cosa non è una riforma in questo ambito? Tutto ciò che agisce parzialmente e contraddittoriamente rispetto ad un disegno unitario e finalizzato; tutto ciò che distrugge o smantella senza prospettare una vera alternativa. Prendiamo il testo in esame, che richiama nel titolo la potestà genitoriale: aiuta la riforma nel suo percorso, ne è una sua anticipazione, o è un alibi per una mancata riforma che rappresenta, in realtà, un arretramento nella tutela dei minori e dei loro diritti? Partiamo già dal titolo: parrebbe occuparsi della potestà genitoriale, ma inganna. Il testo non riforma nel senso di una responsabilità genitoriale, né tanto meno entra in sintonia con le indicazioni europee. Il testo almeno abolisce le odiose e incostituzionali diseguaglianze tra figli legittimi e figli naturali? La risposta è no, e va detto con nettezza. Non c'è una norma, una parola, una riga sulle discriminazioni nei confronti dei figli naturali

come ad esempio in materia di attribuzione del cognome e in materia successoria. Resta tutto immutato, uguale a prima. Quindi, sarebbe mentire veramente a noi stessi affermare che si parificano i diritti tra bambini legittimi e naturali. Ma almeno se ne parifica il trattamento processuale nella crisi della coppia genitoriale? No, anche in questo caso la risposta è negativa. Riguarda in effetti solo i procedimenti relativi alla tutela dei figli nella crisi della coppia, in un modo molto particolare: non prevede che nella crisi della coppia genitoriale non coniugata debba intervenire un giudice a tutela dei diritti dei figli; non prevede nulla per i figli dei genitori naturali che non abbiano mai convissuto; non prevede la possibilità per i genitori, se sono d'accordo, di adire il giudice con un ricorso congiunto, come è possibile nella separazione consensuale; non prevede la possibilità per il giudice di allontanare il genitore non assegnatario dalla casa familiare; non equipara le garanzie; non prevede un rito *ad hoc* come quello della separazione e del divorzio, nei quali i figli dei genitori coniugati ricevano tutela dei loro diritti. Gli stessi provvedimenti provvisori sono lasciati alla discrezionalità del giudice, che può o meno assumerli, mentre è evidente che i figli naturali debbono sapere da subito

non è previsto che i provvedimenti provvisori e definitivi costituiscano titolo esecutivo; non è prevista e disciplinata una fase istruttoria; rimangono i termini giugulatori per l'impugnativa e vi sono limitazioni anche nel ricorso in Cassazione.

in quanto incide solo sul piano del riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, con una logica sostanzialmente punitiva nei confronti del giudice specializzato. che la particolarità della giurisdizione minorile e della famiglia rifugge dalla logica meramente contrappositiva della giurisdizione ordinaria per essere una giurisdizione per la tutela dei diritti nella ricostruzione dei rapporti personali e giuridici su assetti diversi. Non considera che la giurisdizione sulla persona persona e le relazioni familiari pretende un giudice con particolari competenze e attitudini, senza le quali si ha la mortificazione dei diritti e non la loro tutela. Non considera che nella maggior parte dei tribunali non sarebbe possibile prevedere una sezione specializzata per i minori e le relazioni familiari e la materia, con le sue caratteristiche costituzionali e sociali, verrebbe trattata promiscuamente ad altre, con logiche e ricadute sociali completamente diverse. Non considera, infine, il carico ulteriore dei tribunali ordinari - già oberati di competenze - che comporterebbe un incremento inflattivo della giustizia civile

di tutte le altre controversie, in assenza di applicazione di ulteriori risorse, e di dilatare i tempi di giustizia anche nelle controversie che riguardano i minori, per le quali siamo tenuti anche da convenzioni internazionali, oltre che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alla massima tempestività. Serve allora questo provvedimento, o copre un'imbarazzante assenza di progettualità e di scelte di fondo a tutela di soggetti deboli che, proprio per questo, hanno garanzie costituzionali forti?

vogliamo richiamare la responsabilità dei proponenti ad una riflessione e a mettere mano ad una riforma vera. Siamo pronti a confrontarci, e per questo chiediamo di rinviare il disegno di legge

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora relatrice, capisco che il capitolo sul quale si sta soffermando l'attenzione dell'Aula è di straordinaria delicatezza e suscita, com'è ovviamente giusto che sia, un interesse anche emotivo, poiché, come diceva giustamente la relatrice, appartiene ormai compiutamente e in maniera del tutto condivisa alla coscienza di ciascuno di noi la convinzione che non debba esservi discriminazione nel trattamento dei figli illegittimi e dei figli nati fuori del matrimonio.

È ovvio che comunque si tratta di un provvedimento parziale. Ciascuno di noi ha assolutamente presente la bella discussione svoltasi tra i colleghi (dico bella non soltanto perché vi ho partecipato e quindi la ricordo la ricordo con grande piacere, ma anche per la profondità e la qualità della partecipazione) che in dieci anni di discussione tra Camera e Senato hanno esaminato questi temi. piacere il lavoro svolto dalla collega Lussana della Lega Nord nella Commissione giustizia della Camera e ricordo anche quante volte su questi temi ci siamo intrattenuti, nella convinzione che dovessimo arrivare nel più breve tempo possibile ad una riforma di sistema che consentisse a tutti i minori, nati all'interno del matrimonio che quelli nati fuori del matrimonio, di avere un proprio giudice, un giudice specializzato. Ricordo anche il cammino faticoso, che io stessa ho fatto, per arrivare a condividere l'idea del cosiddetto tribunale della famiglia. Qui, guardate, non si discute se tale organo debba essere composto da giudici minorili o da giudici ordinari specializzati, specializzati, quello che importerebbe è che si tratti di un tribunale composto da un giudice specializzato, appositamente formato per giudicare delle molte questioni che riguardano i minori italiani, in qualunque famiglia siano nati:

Questa proposta, da una parte, lasciatemelo dire, elude la questione di fondo. Questo Governo ha ottenuto l'altro giorno una maggioranza molto seria, tanto che tutti gli esponenti della maggioranza continuano a dire che è un Governo nella pienezza della propria forza e che è pronto a fare le riforme; è un Governo che continua a dire che bisogna operare profondamente sui temi della giustizia.

riformina che non elimina le disparità. E perché non le elimina? Lo spiego in due parole. Perché sposta la competenza dal tribunale dei minori al tribunale ordinario, destinandola ad un giudice non specializzato

i figli nati fuori dal matrimonio è prevista una camera di consiglio senza istruttoria, senza garanzia della specializzazione dei giudici. Mi chiedo perché questa disparità.

è vero, un richiamo all'articolo 4 che dice che il procedimento in camera di consiglio senza istruttoria, senza il contraddittorio, che meriterebbe la questione e che potrebbe coinvolgere non soltanto il minore, ma le figure specializzate che devono intervenire in questi casi, deve

Come vedete, rischia di essere una proposta di bandiera che parte da un principio giusto che si perde per strada, ribadendo,

di elaborazione, che ha registrato i nomi non solo di molti colleghi che sono qui, ma anche di altri colleghi. Ricordavo poco fa il contributo della collega Lussana; potrei ricordare ora il contributo del collega Paniz, allora di Forza Italia, che fu determinante. Mi chiedo dunque perché fare oggi una riforma piccola, parziale, che parte da un presupposto giusto ma si perde per strada e, e, purtroppo, si conclude nel sottolineare una disparità e, dunque, nel far registrare al dibattito politico ed istituzionale di questo Paese, rispetto alla frontiera raggiunta, un decisivo, deciso, simbolicamente evidente passo indietro.

Se me lo fa notare persino il senatore Berselli, vuol dire che il livello del cosiddetto brusìo è diventato davvero insopportabile. Come sapete,

Ho ascoltato poc'anzi parole, a giustificare la necessità di rimandare questo provvedimento in Commissione, che fanno riferimento a parzialità e ad incoerenza. difficoltà a comprendere. Mi sono occupato del provvedimento fuori dalla Commissione giustizia, soltanto per una piccola parte. Mi pare che evocare la necessità di una grande riforma, che faccia le cose "più grandi e più belle che pria", sia sicuramente necessario e opportuno. Tuttavia, mi chiedo se rimandare ad una riforma di sistema non rischi di coincidere con un sistema per non riformare, visto che viviamo questo tempo e non un altro. È un tempo in cui non sappiamo bene neanche cosa accadrà di questo Parlamento a settimane e a mesi. Forse, allora, mi porrei questo semplice problema.

insistono nelle ore e nei giorni di ciascuno di noi. È un provvedimento che, mi pare, proprio dallo spirito con cui è stato licenziato dalla Commissione, non voglia opporsi alla possibilità di un'altra, migliore, grande riforma; non mi pare che contraddica o impedisca che quella riforma avvenga. Mi pare che in maniera elementare, perfino con un profilo semplice, tenti di stabilire che il giudice che si occupa della vicenda dei figli nati nel matrimonio sia lo stesso che si occupa dei figli nati fuori dal matrimonio. Non mi pare che È poco? Sì. Serve molto di più? Sì. Serve che questi ragazzi, questi figli, questi «piezz' 'e core» siano francamente uguali in tutto e per tutto. Per adesso possiamo dire questo:

abbiamo sottoscritto il disegno di legge (lo hanno sottoscritto i Capigruppo in Commissione giustizia di tutti i Gruppi, compreso quello del Partito Democratico: sotto questo disegno di legge c'è anche la firma

tale disegno di legge si cerca di andare incontro ad una preoccupazione che esiste nella giurisprudenza e nella dottrina sulla disparità di trattamento a livello processuale tra i figli cosiddetti legittimi, perché nati da due genitori sposati, e i figli nati invece da due genitori che non sono legati dal vincolo matrimoniale. La dottrina più avveduta in materia di diritto di famiglia ci ha segnalato l'opportunità di questa unificazione delle competenze per l'affidamento e il mantenimento economico dei figli, a prescindere dal vincolo giuridico tra i genitori. Dunque è una riforma importante. Certo, non è una grande riforma; prima sentivo parlare della grande riforma del tribunale della famiglia.

basata sul matrimonio e quindi ci sarebbe anche quel problema non indifferente da risolvere. Questo tribunale della famiglia poi cosa fa? Decide sulla famiglia come la prevede la Costituzione o sulla famiglia di fatto, prevista in molti disegni di legge presentati nella passata e nell'attuale legislatura? Dunque, è una riforma intelligente, che va a sanare un problema di conflitto di competenze fra i giudici ed è una riforma che unifica queste competenze, non le separa, e risolve alcuni problemi. Pertanto, chiediamo che ci sia un voto contrario sulla questione sospensiva, che si proceda nell'approvazione del provvedimento, che che ovviamente è stato proposto con questa finalità. Non con la finalità di trovare la soluzione ideale e ottimale nell'assetto giurisdizionale sui delicati problemi dell'affidamento e del mantenimento economico dei figli, ma una soluzione, se volete, anche

Presidente, onorevoli colleghi, quando la presidente Finocchiaro ci ricorda la necessità di una grande riforma della famiglia,

In attesa però che questo si realizzi, bisogna stare fermi? Bisogna conservare la situazione attuale, o vogliamo fare una riforma che (io non dico che sia grande o piccola) è comunque necessaria? Ce lo chiedono tutti gli avvocati di famiglia italiani, nell'interesse dei genitori, ma anche e soprattutto nell'interesse dei figli minori. È un'esigenza

le critiche avanzate dalla senatrice Serafini e dalla presidente Finocchiaro: legittime, sia chiaro, ma sono critiche di merito. In sostanza, si censurano alcuni passi di questo testo, ma

che interessa tutti i bambini, i genitori e i magistrati, il cui orientamento abbiamo cercato di recepire. Il disegno di legge n. 1412 mira invece a semplificare e a rendere più celeri i procedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei minori.

presente anche la senatrice Silvia Della Monica, attuale Capogruppo del Partito Democratico in quella Commissione, che ha condiviso il disegno di legge

Voglio ricordare che la Camera dei deputati in sede legislativa ha approvato all'unanimità il disegno di legge volto a svuotare parzialmente le carceri che stanno scoppiando, prevedendo

Onorevoli colleghi, per cortesia,

Un'occasione mancata, per questo Parlamento, per mettere mano, risolutivamente e definitivamente ad una legge quadro

al fatto di essere ancora - ancora oggi, nel 2010 - considerati bambini legittimi o bambini naturali. È così ancora oggi, nel 2010, dopo che negli

elaborare, e poi ad approvare, provvedimenti e leggi che sicuramente, da questo punto di vista, hanno dato una risposta positiva a questa forte discriminazione. Penso ad esempio alla legge n. 184 del 1983

Proprio in quel momento, proprio 30 anni fa, un gruppo di giuristi - voglio ricordare fra tutti Carlo Alfredo Moro - tentò di mettere mano a quella riforma strutturale a quel tribunale unico della famiglia - con competenze specializzate e con un'adeguata formazione della classe forense che potesse prendere in carico, dal punto di vista giuridico, senza differenziazioni e senza discriminazioni, il problema

non rafforza alcuna tutela e alcuna protezione in favore dei minori. infatti un'equiparazione delle garanzie, non c'è un provvedimento, un punto, un articolo che si prenda cura dell'equilibrio dei minori. Esso non razionalizza il sistema della giustizia, anzi in qualche modo mette in ombra il giudice minorile, e inoltre, voglio dirlo soltanto in un passaggio, non migliora i tempi della giustizia, che in questo modo verrebbero assolutamente peggiorati. L'intenzione sembrerebbe quella di estendere anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati la competenza del giudice ordinario in luogo di quella del tribunale per i minorenni: infatti gli articoli 1 e 2 del disegno di legge mirano a disporre l'abrogazione della disposizione che rimette esclusivamente al padre l'adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili in caso sussista l'incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio l'estensione delle norme sull'affidamento condiviso anche ai figli naturali di genitori che non convivono. Diversamente dai primi due articoli, l'articolo 3 non detta disposizioni sostanziali, ma tende a ridurre le competenze del tribunale dei minorenni in favore dei tribunali ordinari. Dubbi e perplessità solleva la modifica proposta con l'articolo 4 del disegno di legge in esame, intitolato «Disposizioni transitorie», il quale stabilisce che ai processi in corso avanti al tribunale dei minorenni si applichi l'articolo 710 del codice di procedura civile, ovvero lo stesso che a regime andrebbe applicato ai procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori trasferiti al tribunale ordinario. di procedura civile, che affida alla Camera di consiglio la modifica dei provvedimenti della separazione coniugale, è del tutto insufficiente, inadeguato e mantiene, comunque, distinto il rito tra figli legittimi e naturali;

Nei mesi scorsi, insieme ad alcuni colleghi, tra cui i senatori Andria e Mariapia Garavaglia, ho presentato un disegno di legge che persegue la medesima finalità di assicurare il principio dell'eguaglianza dei diritti tra figli legittimi e figli naturali che, pur sancito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, non è stato affermato in modo assoluto, per cui numerose discrepanze persistono nel nostro ordinamento. In particolare, esso interviene a modificare gli istituti della parentela e della successione ereditaria dei figli naturali al fine di eliminare le evidentissime e odiose

La mancanza di una norma che riconosca espressamente tale legame non solo contrasta con il comune sentire - perché è impensabile che un nonno non si senta pienamente e legittimamente tale rispetto ai figli di suo figlio ma anche con altre disposizioni codicistiche, che pure danno rilevanza alla parentela naturale. Il riconoscimento del figlio naturale produce l'effetto di conferire allo stesso uno stato giuridico che lo rende partecipe della famiglia del genitore che lo ha riconosciuto dare un'armonia ed un equilibrio al bambino e alla sua famiglia. Appare, pertanto, davvero doveroso prevedere espressamente questa partecipazione, sancendo il principio che il figlio riconosciuto è senz'altro parente dei parenti del suo genitore. Il riconoscimento dovrà produrre effetti anche nei riguardi dei parenti del genitore che lo effettua, individuando espressamente la parentela naturale come vincolo giuridicamente rilevante anche ai fini successori, con conseguente eliminazione della cosiddetta facoltà di commutazione dell'eredità in

È questa la ragione - lo dico ai pochi colleghi rimasti e alla Presidente - per cui abbiamo chiesto che il provvedimento potesse tornare ad essere

non avrà l'efficacia che si prevedeva potesse avere. Non potrà risolvere neanche questa discriminazione a carico dei bambini: quella di vedere aumentare dolore a dolore, sofferenza a sofferenza, in caso di separazione dei genitori che non sono sposati. La questione andrebbe affrontata diversamente, individuando una riforma organica, costituzionalmente orientata, che ponga sì fine all'insopportabile frammentazione delle competenze giurisdizionali e disciplini compiutamente tutti gli aspetti sostanziali e processuali in tema di famiglia sia legittima che di fatto - dal punto di vista del minore, mediante l'istituzione di un tribunale unico della famiglia con competenze specializzate prevedendo altresì un'adeguata formazione della classe forense, eventualmente istituendo un apposito albo di avvocati specializzati.

Ha chiesto di intervenire la senatrice

Sono convinta, dopo aver ascoltato anche gli interventi delle colleghe della mia parte politica, che esiste un sentire comune su questo argomento, e ciò è molto positivo. Mi sento legittimata ad intervenire perché, nella mia prima legislatura, quella dal 2001 al 2006, sono stata correlatrice, come rappresentante della Commissione infanzia, sul disegno di legge sull'affido condiviso, che oggi è legge.

Anzi, mi permetto di dire che, interpretando chi sta fuori dall'Aula (mi sento infatti espressione di quelle persone, come credo molti di noi), possiamo affermare

persone che purtroppo hanno vissuto una condizione di separazione; purtroppo, siamo tutti a conoscenza dei gravi conflitti

credo che di fronte a questa fotografia

quanto credo che oggi vogliamo affrontare soprattutto quella fattispecie. Chiamiamolo come vogliamo; l'importante è che oggi o domani,

per individuare il giudice specializzato che deve affrontare con competenza e risolvere quei casi che sono risolti in costanza di matrimonio. Mi riferisco alla circostanza in cui i genitori hanno fatto una scelta diversa e i

Interpretando anche il consenso originario che una parte del nostro Gruppo ha espresso, credo che qui, oggi, dobbiamo far uscire una legge diversa da quella che è arrivata in Aula. Mi auguro ci possiamo stringere la mano con senso di responsabilità ed approvare una legge migliore, che risponda davvero a quei bambini,

Signora Presidente, senatrici e senatori, credo che da una parte e dall'altra ci stiamo nascondendo dietro l'ipocrisia, che per certi versi è stata anche palesata poco fa dalla relatrice. Questo disegno di legge, che comunque mi auguro venga approvato, non risolverà le discriminazioni che esistono tra i figli nati dentro e i figli nati fuori dal matrimonio. La discriminazione resterà anche soltanto nei termini:

perché comunque da una parte e dall'altra i riti saranno diversi anche nel caso che sia lo stesso tribunale ad affrontarli;

questo Parlamento in una settimana, un mese o due mesi riesca ad affrontare quello che da decenni non riesce a risolvere, cioè la riforma del diritto di famiglia;

le argomentazioni della senatrice Baio potrebbero essere utilizzate per sostenere la necessità di una legge che vada ad intervenire, per esempio, sulle coppie di fatto, sulle unioni civili. Siamo sicuri che in una settimana siamo in grado di fare una legge sulle coppie di fatto e che ponga fine alla discriminazione dei figli nati dentro e fuori del matrimonio? Siamo sicuri che questo Parlamento, come sosteneva la capogruppo Finocchiaro, sia pronto per affrontare tutti gli argomenti del diritto di famiglia? Le adozioni dei *single*? Siamo davvero pronti? Magari, me lo auguro,

Commissione all'altra, di legislatura in legislatura, ed attualmente è arenato alla Camera, quando nella legislatura scorsa si era arenato al Senato, ma sempre arenato resta? Un argomento in realtà che dovrebbe essere davvero di facile trattazione.

e anche con degli emendamenti, un altro argomento che dovrebbe essere facile da affrontare è la possibilità per i "figli incestuosi" di essere riconosciuti. Siamo in grado di affrontare tutti questi argomenti? Sinceramente me lo augurerei, ma non lo vedo possibile. Allora, a fronte di questo bene, di questa soluzione ottimale del rimettere mano alla riforma del diritto di famiglia, credo che intanto qualche piccolo pezzettino per cercare di eliminare alcune disparità e discriminazioni forse sarebbe anche utile farlo. Faccio un esempio. Quanti di noi per esempio propongono piccoli interventi sulle leggi, piccole modifiche del codice del codice penale o civile? Noi radicali abbiamo depositato tanti piccoli disegni di legge, ma sugli argomenti che citavo prima: l'adozione dei singoli, il divorzio breve, il doppio cognome, i figli incestuosi, i matrimoni *gay*. Poi abbiamo anche depositato un disegno di legge più complessivo: un volume intero che affronta invece *tout court* il diritto di famiglia per una sua revisione completa.

fine di questa discriminazione tra figli legittimi e figli naturali. Vi faccio un esempio: attualmente, ho una figlia naturale; naturale; se invece fossi sposata avrei una figlia legittima. Se io e il mio compagno ci lasciamo, dipende: le cose cambiano se siamo o non siamo sposati.

Grazie se io e il mio compagno risiediamo a Firenze, andiamo al tribunale dei minori, che a Firenze c'è; se siamo residenti ad Arezzo, dobbiamo andare a Firenze. a Firenze. Credo che già questo sia un segnale che ci sia qualcosa che non funziona, perché è evidente che la coppia che si separa, se non è sposata, avrà dei tempi di attesa più lunghi, dovrà spostarsi per accedere al tribunale, dovrà scegliere un avvocato a caso in una città che non è la propria, oppure pagare la trasferta al proprio avvocato locale, o ancora pagare il proprio avvocato e in più l'avvocato domiciliatario. Io credo che questi siano

I tribunali ordinari sono 165, ben più delle Province: i tribunali per i minorenni sono 29, sedi distaccate incluse. È un'argomentazione banale, direte, che interessa soltanto alle coppie? Non credo, perché poi le coppie sono quelle che hanno anche questi

vada avanti. Abbiamo presentato anche due ordini del giorno che sottolineano quello che dicevo all'inizio: certo, non è la riforma del codice della famiglia, si poteva fare di più, si potevano aggiungere altre cose ed eliminare altre discriminazioni che sempre riguardano i figli. Ne abbiamo sottolineate due negli ordini

L'articolo 537, terzo comma, del codice civile prevede un anacronistico e ingiustificato meccanismo dal quale può derivare l'esclusione dei figli naturali dall'eredità e la traduzione del loro diritto in un equivalente economico senza assunzione della qualità di erede. l'articolo 565 c.c., a sua volta, non riconosce un rapporto di parentela tra fratelli naturali. Questa norma è stata oggetto di dichiarazioni di incostituzionalità, ma la Corte Costituzionale, nell'affermare il principio, l'ha modificata solo in parte, sostenendo che compete al legislatore una riforma integrale di essa;

che si esaurisce in questo piccolo nucleo uomo, donna e bambino, o magari due bambini: nel tempo, la società si è data altre forme di organizzazione che la legge italiana non riconosce),

L'altro ordine del giorno che devo illustrare in sede di discussione generale riguarda un argomento, mi verrebbe da dire, tabù o scabroso. Si tratta dell'incesto: ma non per parlare di questo in quanto tale, ma per affrontare il tema di come davvero in questo caso le colpe, anzi in questo caso i peccati, dei genitori ricadono sui figli. I figli incestuosi sono gli unici a cui è negato un un diritto basilare, la possibilità di assumere uno *status* *filiationis*, il diritto ad essere riconosciuti. Altra cosa poi può essere chi avrà la potestà genitoriale, chi se ne dovrà far carico, chi ne dovrà assumere la responsabilità; l'incesto, Ma certo è che quei figli, che non hanno alcuna colpa di essere nati da quei due genitori, sono gli unici che nel nostro codice civile non possono essere riconosciuti, a meno che uno dei due genitori dica che al momento del concepimento non sapeva

credo che questi argomenti sarebbe utile che venissero trattati e affrontati, e mi auguro che anche nel trattare gli ordini del giorno ci sia poi una presa di coscienza che esistono questi casi. Saranno pochi? Non importa, è bene che il nostro codice venga ripulito

Le cose non sono andate, presidente Berselli, come lei ricordava, me lo consenta. In realtà, il Governo aveva annunziato la presentazione del disegno di legge sul tribunale della famiglia; ma dico di più, non soltanto la sottosegretaria Casellati se ne era fatta carico

Grazie

sia per la necessità di un giudice specializzato e continuamente formato, competente per tutta la materia relativa ai diritti della persona, minorenne o adulta, o della famiglia nel suo complesso, legittima o di fatto, con il proposito di abbattere una discriminazione immorale e incostituzionale tra figli legittimi e naturali. Questa volontà condivisa e forte doveva trovare un diverso sbocco. Ecco la ragione per cui oggi insistiamo

in una effettiva parificazione dei diritti dei figli naturali e dei figli legittimi. La disparità che si creerebbe in sede processuale processuale finirebbe con l'incidere ancora di più sotto il profilo discriminatorio sottraendo ad un giudice specializzato, qual è il giudice costituito dal tribunale per i minori, una competenza a favore del tribunale ordinario

di riconoscere al diritto di famiglia e minorile una sua assoluta importanza in una società come quella attuale sempre più complessa, sempre più piena di problemi.

Poiché questa evoluzione non si è compiuta e poiché improvvisamente è stato rimesso in pista un disegno di legge che era stato messo in *stand by*

sono talmente evidenti le ragioni ispiratrici dell'importante modifica al codice civile che andremo ad introdurre con l'approvazione del disegno di legge oggi all'esame del Senato che sembrerebbe superflua qualsiasi disquisizione, dissertazione o considerazione politica sui molti temi sottesi a questo provvedimento: l'eguaglianza di tutti i cittadini, tali solo per il fatto di essere nati, il riconoscimento dell'evoluzione del concetto di famiglia, la massima tutela dovuta dal complesso delle norme ai minori, la necessità di semplificazione, inequivocabilità e velocizzazione dei procedimenti che riguardano la genitorialità genericamente intesa (anche se sarebbe più corretto parlare di bigenitorialità) e vieppiù nei particolari casi di filiazione naturale, di separazione dei coniugi, voglio aggiungere, e in quei rari casi di filiazione incestuosa della quale ancora oggi abbiamo difficoltà a parlare e ragionare. Non credo si debba oggi affrontare il tema di come e se la legge n. 54 del 2006, quella comunemente detta dell'affido condiviso, abbia raggiunto l'obiettivo ambizioso della sua premessa, e cioè «il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi». A quanto afferma la gran parte del mondo forense sembra che ciò non si sia affatto realizzato. Ma è in Commissione giustizia del Senato un disegno di legge su questo tema: ne parleremo, ne discuteremo e comprenderemo le ragioni della disapplicazione, del fallimento o del rilancio dell'affido condiviso. È importante invece che oggi qui, con la modifica degli articoli 316 e 317-*bis* del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso, venga a cessare una sorta di non voluta, ma reale discriminazione su questo tema in relazione ai figli nati fuori del matrimonio. Permangono molti altri temi, quali il riconoscimento del minore, l'attribuzione del cognome, le autorizzazioni per i matrimoni tra minori, la decadenza e la reintegrazione della potestà,

Affermiamo così un fondamentale principio di uguaglianza dei cittadini costituzionalmente garantito; principio di uguaglianza che appare ancora più costitutivo dell'ordine civile quando il soggetto è un minore, un bambino, un figlio, voluto o non voluto, un essere umano, una persona dalla fragile personalità in evoluzione e formazione. Ancor più fragile proprio perché, magari, non ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia tradizionale, quella giustamente sancita e tutelata dall'articolo 29 della nostra Costituzione, quella famiglia in cui non solo ci si può sentire affettivamente, emotivamente e socialmente protetti, ma anche ogni garanzia giuridica è blindata e chiaramente riconosciuta. Le preoccupazioni a suo tempo manifestate dall'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia, in parte recepite, appaiono oggi politicamente superate dall'ampia convergenza su questa legge, che era stata manifestata da tutti i membri della

troviamo oggi qui la sintesi per un intervento che sana un grave *vulnus* del nostro ordinamento, che peraltro ha determinato criticità dovute ai tempi di intervento del tribunale dei minorenni, alle scarse garanzie del rito, ai conflitti e alle parcellizzazioni di competenza. È questa una miniriforma a costo zero, più volta affrontata senza successo in precedenti legislature, che non solo mette fine ad un'intollerabile situazione di incertezza e di giustizia negata, ma che comporta di per sé un decongestionamento dei tempi e dei costi. Saremo così in grado di scongiurare una serie di incidenti processuali in conseguenza del doppio regime, cosi come potrebbero configurarsi a seguito dell'ordinanza n. 8362 del 2007 della Corte di cassazione. Certo è che tutti auspichiamo, come anche il Governo ha più volte annunciato, l'istituzione di un tribunale per la famiglia, unico e a competenza esclusiva per le persone, i minori e la famiglia; una riforma complessa di natura ordinamentale e procedimentale, che, probabilmente, potrà presto inserirsi nel complesso della riforma della giustizia. Una riforma che dovrà necessariamente tener conto dell'esperienza e dell'alta professionalità maturata all'interno del tribunale dei minori, che non realizzi semplicemente una sezione specializzata del tribunale ordinario, ma un tribunale che abbia competenza civile e penale. Una riforma che, partendo dalla Convenzione dei diritti del fanciullo dell'ONU del 1989, riguardi ogni procedimento della persona in età evolutiva. Una riforma che metta al centro l'interesse primario del fanciullo, del minore, che da un lato tenga conto della evoluzione sociale e culturale in atto, che va sbilanciandosi verso il diritto alla libertà dei soggetti adulti, che sperimentano forme di vita familiare sempre più varie e flessibili, ma che dall'altro lato rafforzi la tutela dei soggetti deboli, i minori, che rischiano di uscirne frustrati e penalizzati. Già la Corte costituzionale in prossima successione alla promulgazione della legge di riforma del 2001, in una complessa sentenza, la n. l del 2002, rilevò come non si possa non considerare il minore parte nei procedimenti limitativi e ablativi della potestà (a maggior ragione quando si parla di adottabilità) e quindi ritenere necessario che il minore in questi procedimenti abbia una rappresentanza autonoma dai propri genitori con i quali si trova in conflitto di interessi. Credo che contestualmente vada rimessa al centro dell'azione politica la famiglia, come cellula della società, come luogo di relazioni dinamiche e non somma di diritti e di doveri (grave sarebbe limitarla a questo), come punto di riferimento incrollabile di una stagione infantile, adolescenziale, ma, in realtà, di una vita intera; come istituto giuridicamente tutelato che riproduce nella convivenza stabile del padre, della madre e dei propri figli, paradigmi del diritto naturale; con il ruolo fondamentale dei nonni, ancor più importanti nei casi di filiazione naturale e di genitori separati, dei quali di qui a breve parleremo quando il disegno di legge di modifica sul diritto di visita, attualmente in Commissione giustizia, arriverà in Aula. Eppure in questi ultimi decenni moltissimo è stato fatto: si è voluto restituire dignità ad ogni *status* che potesse apparire socialmente debole o discriminabile, nella sostanza e nella forma, *verba sunt Così come per esempio in tema di lavoro non più spazzini o domestici, ma operatori ecologici e colf, in tema di disabilità non più ciechi o sordi, ma non vedenti o non udenti e comunque diversamente abili, così in tema di filiazione non più figli illegittimi, ma figli naturali, come introdotto dalla riforma del 1975. Ma l'Italia che oggi fotografiamo - mi rifaccio a quanto ha affermato in conclusione la relatrice è assai lontana da quella magistralmente interpretata da Marcello Matroianni e Sofia Loren in «Matrimonio all'italiana» e non è nemmeno quella che sceglie la figlia naturale del più popolare cantante degli anni '60 come *testimonial* di uno *status* e di una possibile rivalsa. Al legislatore non è dato prevenire i fenomeni sociali ma fotografarli e, non appena il fotogramma è passato, fotografarli ancora per correggere, come in questo caso, gli errori fatti. L'Italia che dovremo andare a fotografare a breve, con nuove norme e tutele, è quella delle famiglie allargate o multietniche, che si confronta con nuove povertà di genitori separati, se è vero che il sindaco di Roma ha inaugurato una casa di accoglienza per padri separati indigenti; è quella realtà, e concludo, che sempre più farà i conti con il progresso della scienza e della bioetica che va ben oltre il test del DNA e apre nuove pericolose frontiere e nuove problematiche che gravano sulla famiglia, sull'essere genitori o madri e padri, che forse è ancor diverso, e sull'essere compiutamente figli.

la giustizia*. Signora Presidente, signori senatori, negli ultimi anni l'evoluzione del costume sociale ha determinato notevoli mutamenti: penso all'immigrazione e alla globalizzazione. Anche la famiglia è cambiata e sta ancora cambiando: penso ai giovani e al loro modo di rapportarsi con gli adulti. Famiglie e minori quindi sono stati investiti negli ultimi decenni da mutazioni e cambiamenti radicali. L'aumento delle separazioni e dei divorzi, il crescente numero di matrimoni tra persone di diversa nazionalità, il diffondersi del nuovo istituto dell'affidamento familiare, la riforma del codice civile in materia di affidamento condiviso della prole stanno delineando nuove questioni in tema di famiglia, in cui è inevitabile una nuova sensibilità per le problematiche che attengono ai minori e ai loro diritti. Tutto questo non può non trovare un quadro di riferimento, non solo giudiziario, capace di assistere e promuovere i diritti della famiglia, diritti dei suoi componenti, con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti. Di fronte a tali mutamenti la famiglia e i minori hanno oggi in Italia un quadro di riferimento nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria assai frammentato. La proposta legislativa oggi in esame è frutto di un lavoro parlamentare attento, approfondito, competente svolto dalla Commissione giustizia, e mira a risolvere il problema della inaccettabile parcellizzazione delle competenze fra il tribunale dei minori e il tribunale ordinario nei procedimenti relativi all'affidamento dei figli; parcellizzazione che è fondata unicamente sulla diversa qualificazione dei soggetti coinvolti quali figlio nato all'interno o al di fuori del matrimonio. Ed è questa la vera disparità. È questa la vera discriminazione. È un provvedimento che afferma con forza il principio in virtù del quale tutti i figli minori, siano essi i figli naturali o i figli legittimi, devono avere la stessa tutela, la più ampia, equa e profonda possibile, sul presupposto che la condizione giuridica dei genitori in relazione al vincolo coniugale non può determinare una condizione diversa, non può determinare differenze nel trattamento giuridico dei figli. Devo sottolineare che l'approvazione di questo provvedimento costituisce un primo passo importante nella direzione di una più generale unificazione della materia, come ha sottolineato del resto la senatrice Gallone, che da un punto di vista processuale dà anche ampie garanzie di contraddittorio e quindi ampie tutele. È per questo che ne auspico l'approvazione. Ritengo - l'ho detto più volte anche in Commissione giustizia - che questo provvedimento sia solo anticipatorio di una più completa e generale sistemazione della disciplina, che si potrà realizzare solo attraverso il disegno di legge allo studio del Governo che istituirà il tribunale della famiglia. Questo nuovo istituto, che si avvarrà, lo ripeto ancora, di giudici, avvocati specializzati, esperti in una disciplina che richiede sempre conoscenze specifiche e sensibilità, Il nuovo istituto costituirà poi ciò che è stato richiesto da più parti con voce forte, decisa, vale a dire quel terreno utile a superare quella che anche noi consideriamo l'anacronistica disciplina dei diversi *status* di figlio legittimo e naturale; disciplina che caratterizza purtroppo ancora oggi, del tutto inopinatamente, l'ordinamento giuridico italiano. È stato sottolineato più volte, e lo pensiamo anche noi con forza, che i figli devono essere uguali, i figli non devono avere aggettivazioni e nessuna discriminazione. I figli sono figli e basta.

di Bruxelles II del 2003 che segnala l'esigenza di abbandonare il termine potestà per definire il rapporto tra genitori e figli, sostituendolo con quello di responsabilità genitoriale. È evidente infatti che, mentre il primo sottolinea i diritti degli adulti, il secondo mette in evidenza i loro doveri nei confronti della prole. È anzi da notare che l'emendamento interviene nel modo più sobrio possibile, evitando di sostituire un termine con l'altro - come sarebbe stato più rigoroso fare - ma limitandosi ad affiancare il secondo al primo, proprio con l'intenzione di restare il più aderenti possibili alla formulazione originaria. L'adeguamento, d'altra parte, trova la sua prima e immediata applicazione con l'emendamento al testo che sottolinea la nuova ottica nella relazione tra figli e genitori, assicurando ai primi il mantenimento di una doppia protezione anche dopo la rottura del legame di coppia fra i genitori. Si tratta dunque, per quest'emendamento, come per gli altri,

È questo il motivo, ad esempio, per il quale il termine "cura" è stato separato dagli altri tre di cui all'articolo 30 della Costituzione. L'assegnazione di compiti di cura a ciascun genitore, infatti, è esattamente la modalità che realizza il cambiamento rispetto al passato, in cui un genitore poteva liberare se stesso da ogni incombenza accontentandosi accontentandosi di dare del denaro all'altro affinché quest'ultimo provvedesse ad ogni necessità dei figli. Spesso questo ruolo lo ricopriva l'uomo: il marito versava - e versa tuttora - l'assegno mensile alla donna, alla madre, che prende i soldi donna, alla madre, che prende i soldi ma poi, per altri versi, assolve a tutti i compiti. L'ultimo emendamento, infine, approfitta dell'occasione di mettere mano al diritto di famiglia per correggere un'evidente e grave stortura dell'attuale formulazione in riferimento all'interesse morale e materiale della prole. Infatti ha senso ed è indispensabile proprio quando la norma, riferendosi genericamente ad altre decisioni, lascia il giudice privo di un criterio che le ispiri. Come è ben noto, non è la prescrizione diretta, come l'affidamento condiviso, definito da specifiche norme di una legge *ad hoc*, ad avere bisogno di una guida per l'applicazione, ma ciò che residua, che non è esplicitamente normato e che fa riferimento soltanto a principi di carattere del tutto generale.

sottolineare al presidente Berselli, alla relatrice e al Governo che l'abbassamento dell'età a 12 anni

da genitori non coniugati e aderire - assumendo la regola valida

Mi spiego: si tratta di due istituti completamente diversi, perché da un lato si parla di minori che abbiano compiuto 12 anni o che abbiano un'età anche inferiore ove capaci di discernimento, ma lo si fa in materia di separazione.

e ciò ha fatto sorgere dubbi applicativi con gravi ricadute sul fatto che le disposizioni introdotte dalla legge n. 54 del 2006, la cosiddetta legge sull'affido condiviso, si possano applicare anche alle coppie che non abbiano mai convissuto. Poiché non vorremo questo, ecco la ragione di questo emendamento. Inoltre, con l'emendamento in esame si vogliono applicare istituti e garanzie previsti a tutela del genitore debole al quale non sia addebitabile la separazione

cosa che è particolarmente importante quando i procedimenti sono definiti con decreto che altrimenti non darebbe una possibilità di iscrizione di ipoteca giudiziale e del pagamento diretto (comma Non è sufficiente purtroppo estendere questi istituti e garanzie previsti dall'articolo 156 del codice civile ai casi dei figli di genitori non coniugati in quanto compatibili poiché la norma si riferisce di base esplicitamente ai soli coniugi

ordinario. Per le ragioni che abbiamo già esposto, non è condivisibile la scelta di operare una riforma criptica di carattere ordinamentale, che finisce con l'erodere la competenza del tribunale per i minorenni semplicemente

civile, riferito alla condotta dei genitori pregiudizievole ai figli e, nello specifico, all'allontanamento di un genitore, che riteniamo sia opportuno venga contestualizzato, anche se la questione interviene in sede di separazione in corso. È corretto, quindi, che in tal caso la competenza rimanga al tribunale ordinario.

Grazie abbiamo ascoltato molte delle ragioni espresse dai colleghi del PD ci si rende conto che questo è un provvedimento che non può affrontare - e non voleva farlo - molti degli altri aspetti, pur validamente esposti e meritevoli di approfondimento.

con acutezza indicato nell'ultimo periodo della sua relazione. Viene così a cessare l'ingiustificata duplicazione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni fondata unicamente sulla diversa qualificazione di uno dei soggetti coinvolti quale figlio nato all'interno, o al di fuori, del matrimonio. In fondo, il cuore del provvedimento che noi stiamo votando è proprio questo. I ragionamenti che abbiamo svolto in Commissione andavano in questa direzione. Speriamo di poter in seguito approvare altri provvedimenti che seguono questa linea. Votiamo convintamente questo provvedimento considerandolo anche un auspicio di una riforma più radicale.

incoerenza tra le molte, una contraddizione tra le molte, senza impedire che le altre molte contraddizioni ed incoerenze vengano successivamente risolte. Votiamo questo provvedimento perché è leale ed affronta e risolve subito quel che può, sapendo che quel che si dovrebbe fare, fare, come è stato opportunamente elencato dalla senatrice Poretti - cui riconosco da sempre peraltro una straordinaria onestà intellettuale - non è né semplice né immediato poter affrontare. Votiamo favorevolmente perché ogni buona legge ha in sé un piccolo contenuto pedagogico-culturale: ed anche questa lo ha. Sostanzialmente, dice che davvero l'affidamento condiviso diventa un po' più uguale per tutti, e quel termine uguaglianza dovrebbe pur dare qualche suggestione particolare. Certamente la dà a noi che da sempre, nei figli, in tutti i figli,

Signor Presidente, riconfermiamo il nostro voto positivo a questo provvedimento che, come è stato detto, consente di fare un passo avanti nella tutela dei figli naturali. Oggi possiamo dire che c'è e ci sarà, con l'approvazione di questo provvedimento, un'equiparazione della posizione dei figli naturali a quella dei figli legittimi, quantomeno sotto il profilo processuale della competenza giudiziaria. Serve ancora un cammino verso una parificazione sotto il profilo di diritto sostanziale, ma con questo provvedimento un obiettivo importante, di parificazione sotto il profilo processuale, possiamo dire che sia raggiunto. È un obiettivo che il mio movimento, la Lega Nord, ha perseguito anche negli anni passati.

vedo che c'è molta fretta di concludere i nostri lavori. Noi non ci opporremo certamente, non facciamo ostruzionismo; ma vogliamo essere chiari, per evitare equivoci. Ritengo sia quanto mai singolare che nel nostro Paese non si riesca a mettere d'accordo le forze politiche neppure quando si trattano argomenti il cui contenuto, la cui essenza, non solo non le trova distanti ma addirittura le vede convergenti. È stato detto in maniera chiara quanto siamo d'accordo, quanto siamo convinti; anzi, abbiamo alle spalle la prova storica del nostro impegno diretto a garantire un principio sacrosanto e costituzionale quale quello della parità di trattamento, dell'uguaglianza dello stato giuridico, che bisogna riconoscere a tutti i figli, senza distinzione alcuna. Allora, perché questo contrasto che è emerso in Aula? Perché noi riteniamo che questo disegno di legge non sia coerente con le finalità e con gli scopi che hanno presieduto alla sua presentazione. Dice il collega Berselli che la firma dei rappresentanti dei vari Gruppi - quindi anche del nostro - renderebbe la nostra posizione critica quale oggi è, incoerente e quindi inaccettabile. Non è così, non è questa la realtà dei fatti. L'assenso del nostro Capogruppo del momento fu dato in un contesto ben differente, in cui eravamo sicuri e certi che si trattasse di un disegno di legge che voleva

l'intenzione e il programma concreto del Governo di presentare un disegno di legge risolutivo - almeno noi ci auguriamo che possa esserlo - di tutti i problemi che attengono nel complesso

che posso definire abbastanza concorde, sia pure con una certa dialettica, all'interno della nostra Commissione, e poi c'è stata una evoluzione che è stata tratteggiata in maniera precisa, e inconfutata, dalla collega Della Monica. Lo stesso Governo ha segnalato - ed è stato apparentemente seguito - la necessità e l'opportunità di rallentare l'attività della Commissione, o comunque l'attività relativa all'esaurimento della procedura normativa riguardante il disegno di legge che ci apprestiamo a votare. Perchè tutto questo? Per le ragioni che la stessa sottosegretaria Alberti Casellati ha oggi illustrato e che io richiamerò alla fine di questo mio breve intervento. Noi critichiamo in maniera convinta questo disegno di legge perché parte con l'intenzione dichiarata di voler favorire favorire il rispetto del principio di uguaglianza tra i figli legittimi e naturali, e invece non lo fa; addirittura, noi riteniamo che la situazione vada a comprometteresi ulteriormente. Non lo fa perché non tocca i principi essenziali, i punti nevralgici, tutti nevralgici, tutti quei temi che la collega Serafini ha elencato e che non sto qui a ripetere, ma che in maniera succinta richiamo: i problemi della casa, dell'assegnazione della casa nel rapporto di coppia quando non si ha davanti una famiglia legittima;

Cosa affronta allora? Affronta il problema della competenza. E qui riemerge a mio giudizio una tendenza che nel centrodestra si è manifestata in maniera pericolosa, devo dire neutralizzata da alcune forze dello stesso centrodestra, quando c'è stato un tentativo di cancellare dal nostro sistema giuridico i tribunali per i minori. Sto parlando di uno dei punti di eccellenza del nostro sistema giuridico e giudiziario, di uno dei pochissimi giudici specializzati che nascono con la nascita del diritto minorile in Italia, frutto di battaglie e di impegni culturali e giuridici che hanno dato al nostro Paese quello che è un vanto e che viene preso in considerazione e anche a modello da moltissimi Paesi civili ed

un fervore di trasformazioni delle quali bisogna tener conto perché questi fenomeni incidono sull'istituto della famiglia. Siamo d'accordo, ma è questo il motivo per cui ci siamo acquietati, questa la ragione per cui avevamo fiducia in quella che, se se non è un impegno formale, signora Sottosegretario, era un dichiarazione di intenti, e noi puntavamo a questo. Noi sentiamo che almeno da parte della Sottosegretaria c'è questa posizione che equivale alla nostra; non era e non sarebbe necessario, se non lo volessero alcuni di voi, andare alla ricerca disperata ed affannosa in questo momento di esibire qualcosa a tutti i costi. È difficile, lo riconosco, spiegare ad un'opinione pubblica, che attende riforme vere e serie, perché noi oggi diremo di no ad un disegno di legge di questo tipo. Non vogliamo forse che i figli naturali minori siano equiparati ai figli legittimi? Non è vero, tutto questo. Noi avremmo voluto

la vera riforma che mette in condizione un sistema giudiziario di funzionare, la vera riforma che dia dignità a questi soggetti che hanno bisogno di riconoscimento dei diritti, non verrà mai. Cosa fa questo disegno di legge? Frammenta Non raggiungete nessun obiettivo, e la ragione è chiara: volete esibire, non so in quale sede, forse in un'immaginaria ma non troppo lontana sede elettorale, di avere tirato fuori anche un nobile documento legislativo a favore dei figli naturali. che questo non sia corretto e leale dal punto di vista istituzionale. Comunque, prendiamo atto della dichiarazione della Sottosegretaria, che sostanzialmente non smentisce la ricostruzione fatta dalla collega Della Monica e dice che il Governo è ancora intenzionato, il Governo seriamente vuole porre mano alla riforma, che poi non sarebbe tanto difficile e lunga. Quindi, non capisco perché questo atteggiamento di sfiducia da parte di una maggioranza ancora così forte, almeno formalmente, rispetto a disegni di legge che potrebbero veramente essere utili al Paese. Prendiamo pertanto atto delle dichiarazioni di intenti della Sottosegretaria per la giustizia, che oggi ci viene a ribadire l'interesse serio e concreto del Governo a presentare una riforma che preveda il tribunale per la famiglia: un tribunale quindi che, se mai si dovrà vedere, non sostituisce il tribunale per i minorenni ma lo integra, lo sviluppa, lo rende più completo, cioè un giudice altamente specializzato. In considerazione di ciò e volendo offrire una nostra posizione critica costruttiva, noi non voteremo contro ma ci asterremo nella votazione di questo disegno di legge. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, si è parlato in questa Aula di un'occasione mancata: mancata: sì, colleghi del Gruppo del Partito Democratico, un'occasione mancata, ma sicuramente non per responsabilità dei presentatori di questo disegno di legge; sicuramente non per responsabilità dei componenti

Esordendo, la senatrice Gallone aveva fatto riferimento al fatto che oggi avremmo potuto scrivere tutti insieme una non rara, ma certamente infrequente bella pagina di storia parlamentare, che noi oggi non scriveremo. Non la scriveremo perché improvvisamente, con una sorta di rivoluzione copernicana del vostro percorso, colleghi del Partito Democratico, introducendo tra l'altro una categoria assolutamente inusuale

all'unanimità, nella Commissione fisiologicamente deputata, più di ogni altra, ad occuparsi di questioni di diritto, l'avevate integralmente condivisa, al punto che il vostro Capogruppo dell'epoca risulta firmatario di questo disegno di legge),

tacendone peraltro (e tacendo anche a voi stessi) i lunghi ed incerti tempi di realizzazione, le grandi difficoltà per le quali ed è la cartina di tornasole più convincente di questo ragionamento - ancora, nonostante l'intendimento di tutti, non è stata realizzata. Questo disegno di legge non ha la pretesa - non l'ha mai avuta - di essere una grande riforma, ma certamente (questo sì, onorevoli colleghi) è un primo significativo passo avanti verso quella riforma nel solco condiviso da tutti (non c'è stato un intervento che questi principi fondanti non abbia richiamato) del principio della bigenitorialità, dell'equiparazione tra figli legittimi e naturali, della *reductio ad unum* per quanto concerne il giudice naturale dei minori, della necessaria ridefinizione, comunque demandata allo Stato quantomeno delle competenze di quel tribunale per i minorenni che continua ad esistere e che sicuramente non è possibile cancellare *tout con un colpo di spugna, ma che comunque, necessariamente, deve essere in qualche modo rivisitato. Questo complesso di norme non risolve tutti i problemi delicati, complessi ed articolati della tutela dei minori, legittimi o illegittimi che siano, sotto il profilo del rapporto di filiazione, ma alcuni li risolve con assoluta certezza. Lo avevamo compreso perfettamente tutti in Commissione giustizia, avevamo addirittura pensato sede deliberante; poi abbiamo ritenuto di investire tutta l'Assemblea perché ritenevamo che comunque, come i colleghi hanno opportunamente colto, con la logica, se volete, assolutamente prosaica - attingiamo qualche volta alla saggezza popolare - del bicchiere mezzo pieno o dell'ottimo che è nemico del bene nemico del bene potessimo fare un primo significativo passo in avanti. E allora, perché non compierlo insieme, oggi, questo primo significativo passo in avanti? Spiace, colleghi del Partito Democratico - lo dico sinceramente al di là di tutta la pindarica arrampicata sugli specchi fatta in questa Aula - che abbiate cambiato idea. Noi non l'abbiamo cambiata, e questo primo significativo passo lo compiremo insieme a quanti in questa Aula, con senso di realismo e responsabilità, vogliono porre un altro mattone fondamentale della costruzione futura che sarà quell'organica riforma verso la quale questo disegno di legge inequivocabilmente si dirige. Esprimo quindi il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.

Salutiamo con favore l'impegno assunto dalla maggioranza e dal Governo sulla fine della discriminazione, per esempio, in materia ereditaria tra figli naturali e figli legittimi e sulla possibilità che i figli incestuosi possano essere riconosciuti.

*Il Senato approva Pertanto, come stabilito della Conferenza dei Capigruppo, la seduta antimeridiana di domani non avrà luogo, anche al fine di consentire più ampi spazi di lavoro alle Commissioni, impegnate in particolare nell'esame del documento recante la Decisione di finanza pubblica.

alla consigliera nazionale di parità Alessandra Servidori, raggiunta oggi da una lettera di minacce nell'ambito della sua attività, legata anche alla promozione dell'occupazione femminile. La partecipazione femminile al mercato del lavoro è il tema principale attorno al quale si sviluppa l'attività della consigliera nazionale di parità, così come previsto da una famosa legge, forse una delle leggi più importanti dedicate alla parità,

particolare allo sviluppo dell'occupazione femminile. Il ruolo e il lavoro di Alessandra Servidori sono noti a tutti. Da molti anni vive scortata a causa della sua attività intellettuale, innanzitutto come docente.

diversi riformisti, che, nell'ambito del centrodestra, in particolare, ma anche del centrosinistra, si sono spesso trovati raccolti attorno all'idea di modernizzazione del mercato del lavoro.

a non piegarsi di fronte alle minacce; così come ci auguriamo che l'intero mondo del lavoro, nelle parti sociali, nelle categorie, nel sistema più ampio e complesso delle relazioni industriali, possa trovare sempre vicino a sé le istituzioni pubbliche e la politica, per non sentirsi mai abbandonato. Gli episodi di violenza verbale, ma forse anche fisica, continuano a ripetersi. Mi auguro che da nessuno possa venire complicità, anche indiretta e involontaria, a chi pensa di poter intimidire e intimorire il difficile lavoro dei riformisti che, soprattutto nel Governo Berlusconi, cercano di portare avanti le istanze che, invece, spesso nel passato sono rimaste insabbiate nei cassetti, fermate da quel blocco ideologico, che ancora alberga soprattutto in una parte della nostra sinistra e che ha impedito la modernizzazione del nostro sistema. Grazie ad Alessandra Servidori per il lavoro che fa e che continuerà a fare. abbiamo appena ascoltato dalla collega Bonfrisco la notizia di un atto di intimidazione nei confronti di Alessandra Servidori, la quale è conosciuta per il suo impegno a favore dei diritti delle donne e del lavoro. Collega Bonfrisco,

Non ho visto le agenzie, ma non abbiamo motivo di dubitarne. Siamo molto preoccupati anche noi, perché un conto è dibattere, a partire dalle proprie convinzioni, le grandi questione del lavoro,

e sosteniamo Alessandra Servidori in tutte le sue manifestazioni di pensiero e in tutte le sue gesta a favore del lavoro e dei diritti delle donne.

Grazie nella seduta del 2 febbraio 2010, di acquisire della documentazione e dei plichi contenenti schede pervenute da sezioni della ripartizione America settentrionale e centrale, perché vi erano delle segnalazioni, pervenute attraverso dei procedimenti penali, che concernevano dei brogli elettorali pesantissimi nei quali potrebbero essere coinvolti esponenti dei clan calabresi, tra cui il clan Piromalli; si tratta di intercettazioni che erano state acquisite agli atti di un dibattimento. Quindi si chiedeva e si chiede ancora, per l'interesse diretto che ha, oltre che per l'integrità di questo organo costituzionale, anche per gli accertamenti che sta svolgendo la Giunta, di sapere dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno se corrispondano a verità queste segnalazioni sui comportamenti di clan calabresi nell'ambito dei brogli elettorali che hanno colpito la circoscrizione Estero, in particolare in America settentrionale e centrale, e se siano in corso indagini o se siano state effettuate indagini di carattere amministrativo o di polizia giudiziaria concernenti la regolarità delle elezioni del 2008 per questa circoscrizione Estero.

indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze, a proposito di una vertenza tra la ditta Cofiloc Spa e l'Agenzia delle entrate di Treviso. La questione è abbastanza urgente perché il tribunale di Treviso ha rinviato l'udienza in quanto sta aspettando la risposta del Ministero, nel senso che il Ministero deve soltanto confermare la posizione che ha già assunto il il 23 maggio 1996, a seguito anche della sentenza della Corte di cassazione n. 13506 dell'11 giugno 2009, dove si dice che il criterio sostanziale deve essere ritenuto conforme allo spirito del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, in riferimento alla errata interpretazione della tabella dei coefficienti di ammortamento nel bilancio di questa ditta.

17 giugno 2010. Questa interrogazione ha come oggetto il finanziamento per i terremoti avvenuti in Umbria nel 2010. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento mi ha fatto sapere di aver inoltrato ai Ministri competenti la sollecitazione che la Presidenza del Senato gli ha fatto

Nell'impazzare di agenzie, di commenti del Governo, di senatori, deputati e quant'altro, credo che il Parlamento forse dovrebbe essere coinvolto sull'argomento.